aperta la votazione.

L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 26 settembre 2013.

Questa settimana, dopo la discussione dei disegni di legge di rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato si passerà alle dichiarazioni di urgenza sui disegni di legge segnalati dai Gruppi ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, nonché all'esame della Relazione governativa sugli effetti per la finanza pubblica derivanti dalle misure contenute nel decreto-legge n. 102 in materia di IMU. Domani mattina, alle ore 11, il Ministro della giustizia renderà un'informativa sulla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, mentre nel pomeriggio, alle ore 16, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà un'informativa sul vertice G20 di San Pietroburgo. Per entrambe le informative i Gruppi potranno intervenire per dieci minuti. Il calendario della settimana corrente prevede infine la discussione di mozioni sulla combustione di rifiuti nei cementifici. La prossima settimana, a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 17, saranno discussi il decreto-legge in materia di valorizzazione dei beni e attività culturali e la ratifica dell'Accordo tra Albania, Grecia e Italia sul progetto «Trans Adriatic Pipeline». Nella seduta pomeridiana di mercoledì 18 si procederà alla votazione per l'elezione di due componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria. D'intesa con la Presidenza della Camera dei deputati, si procederà alla convocazione per la costituzione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni bicamerali e delle Delegazioni italiane presso le Assemblee parlamentari internazionali. Giovedì 19, alle ore 16, il Ministro della difesa risponderà ad interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento. Nella settimana dal 24 al 26 settembre l'Assemblea esaminerà il decreto-legge sulla pubblica amministrazione, il Documento istitutivo di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti di amministratori locali, nonché il disegno di legge in materia di demolizione di opere abusive. In apertura delle sedute pomeridiane di martedì 17, mercoledì 18, martedì 24 e mercoledì 25 settembre, saranno ricordate, rispettivamente, le figure dei senatori Giulio Andreotti, Franca Rame, Emilio Colombo e Umberto Carpi.

7 aprile 2011, n. 39, che ha ampiamente semplificato e razionalizzato il complesso delle procedure che presiedono le decisioni di finanza pubblica. In tale contesto, ai fini di un'ordinata gestione finanziaria dello Stato, la legge n. 196 del 2009 ha affidato al rendiconto generale dello Stato il compito di rendicontare al Parlamento, nella forma della legge, l'avvenuto rispetto di quanto autorizzato con la legge di bilancio. Sul piano procedurale e tecnico contabile, la proposta di bilancio a legislazione vigente per l'esercizio 2014, che il Senato esaminerà a partire dal 15 ottobre prossimo, assumerà quale base di riferimento le risultanze definitive contenute nel rendiconto, le quali sono state altresì evidenziate nel disegno di legge di assestamento per il 2013, ai fini della determinazione degli eventuali adeguamenti delle autorizzazioni di pagamento. Il rendiconto, come il bilancio, è articolato in missioni e programmi ed è composto dal conto consuntivo del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite previste dal bilancio dello Stato dell'anno precedente, e dal conto consuntivo del patrimonio, Una novità particolarmente rilevante per il consuntivo 2012 è rappresentata dalla dematerializzazione del rendiconto generale dello Stato, realizzata, per il primo anno, in via sperimentale, di concerto con la Corte dei conti, Inoltre, sul versante del potenziamento dei sistemi conoscitivi va rilevato che anche per il 2012 si è data attuazione alla previsione della stessa legge n.196 circa il rafforzamento del ruolo delle rilevazioni economiche. del bilancio è articolato in missioni e programmi; le missioni sono state 34; il numero dei programmi si è confermato in 172, e nella quasi totalità, essi sono da ricondurre a specifici interventi di ciascuna amministrazione, essendo limitati a soli quattro i programmi condivisi da più Dicasteri. Nel rendiconto 2012 trova conferma l'adozione del nuovo impianto delle note preliminari e la compilazione delle note integrative al consuntivo, che rappresenta la naturale conclusione del ciclo di programmazione e costituisce lo strumento per rafforzare la trasparenza e la capacità delle amministrazioni di rendere conto della propria gestione. Tuttavia, per quanto concerne gli indicatori di *performance* delle amministrazioni, appare del tutto evidente che gli stessi debbano essere ulteriormente rafforzati ed affinati, al fine di dar conto al Parlamento, in maniera più convincente, della effettiva capacità delle amministrazioni di conseguire gli obiettivi loro assegnati attraverso un utilizzo efficiente delle risorse.

Per effetto del varie manovre approvate negli ultimi due anni, l'esercizio trascorso ha evidenziato inoltre una nuova riduzione dell'indebitamento anche rispetto ai due esercizi precedenti, segnando un valore pari al 3 per Il saldo primario in rapporto al PIL si è attestato su di un valore notevolmente in progresso, con un valore positivo pari al 2,5 per cento del PIL. Tali dati evidenziano come le manovre adottate per la correzione dei conti pubblici siano state particolarmente pesanti, con riflessi negativi sulla produzione del reddito, ma necessarie al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede di Unione europea e alla conseguente recente uscita del nostro Paese dalla procedura di infrazione aperta nell'anno 2009. Nel merito, passando ai dati complessivi del bilancio dello Stato, in relazione alle entrate finali, si rileva che gli accertamenti sono ammontati a circa 545 miliardi (in aumento rispetto al 2011), mentre le spese finali si sono attestate a 535 miliardi (anch'esse in aumento rispetto al 2011). Il saldo netto è positivo per circa 10,8 miliardi di euro, dopo che anche nel 2011 si era registrato un saldo positivo, Passando ad analizzare gli altri saldi, si evidenzia l'ulteriore miglioramento del risparmio pubblico, che passa dai 46,1 miliardi del 2011 ai 48,5 miliardi Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario, quale saldo scaturente dal confronto tra il totale delle entrate finali e il totale delle spese complessive, mostra un risultato, per il 2012, che si attesta a 203,5 miliardi di euro, in aumento rispetto al 2011. Nel confronto con i dati gestionali, lo scostamento registrato, per quanto riguarda le entrate finali, tra previsioni definitive e il volume accertato, è stato pari ad un aumento di 9 miliardi, mentre l'omologo dato relativo al 2011 era pari Particolare interesse rivestono le informazioni deducibili dai dati ricavati dall'analisi economica delle spese finali. Al riguardo, è possibile osservare come la spesa di parte corrente abbia generato impegni per 489 miliardi (in crescita rispetto al 2011), mentre quella in conto capitale per circa 45 miliardi (in calo rispetto al 2011),

I dati appena richiamati, pur in un contesto generale di netto miglioramento degli indicatori di finanza pubblica, confermano la difficoltà incontrata nel ridurre e tenere sotto controllo la spesa corrente, che spesso viene compensata attraverso riduzioni ingenti delle spese in conto capitale, che come è noto rappresentano un fondamentale volano per la crescita economica del Paese. La caduta della spesa in conto capitale è il vero dato dolente del rendiconto 2012 riguarda sia i pagamenti sia i trasferimenti in conto capitale alle imprese. Dati preoccupanti si registrano anche con riguardo ai trasferimenti agli enti pubblici e in particolare alle amministrazioni locali, titolari di circa il 70 per cento degli investimenti pubblici, che non a caso denunciano una flessione insostenibile in tale contesto. Passando alla gestione di cassa, limitando l'analisi solo ai saldi, si osserva che nel 2012 il risparmio pubblico al lordo delle regolazioni contabili è stato negativo per circa 19,1 miliardi di euro, in miglioramento rispetto al 2011.

Dalla ricognizione della consistenza dei residui passivi di nuova formazione al 31 dicembre 2012, sulla base della tabella 17 della relazione al disegno di legge, si osserva che circa il 66

Passando all'analisi delle criticità più rilevanti del rendiconto 2012, quelle che destano maggiori preoccupazioni riguardano la trasparenza della rappresentazione di entrate e di spese, il perdurante fenomeno dei residui attivi e passivi e le regolazioni contabili e debitorie: che evidenziano problemi di ricostruzione del bilancio. Come per gli altri anni, anche per il 2012 la Corte dei conti ha sollevato un problema generale di grande rilievo che attiene alla rappresentazione di entrate e spese secondo la contabilità nazionale, come richiesto in sede europea, che presenta difformità talvolta rilevanti rispetto al rendiconto oggetto della parificazione. Per quanto concerne il versante delle entrate, in particolare, l'esame ha confermato la presenza di una serie di elementi contabili incongrui, riconducibili alla categoria delle incongruenze propriamente dette, come importi con segno negativo per riscossioni residui, resti da versare e resti da riscuotere, come conseguenza di accertamenti inferiori alle riscossioni e di riscossioni inferiori ai versamenti, ovvero in anomalie interne al rendiconto, quali l'emersione per una serie di voci di bilancio di insussistenze o di riaccertamenti, cioè di sopravvenienze passive o attive. Nel dettaglio la Corte dei conti ha rilevato l'esistenza di poste di bilancio, riportate in appositi allegati alla decisione, per le quali si sono riscontrate sensibili discordanze dei relativi importi rispetto a quelli risultanti nelle contabilità delle amministrazioni, nonché, in merito alla contabilizzazione nel «riscosso residui» dell'anno, capitoli per i quali gli importi dei residui attivi finali registrati nel rendiconto risultano diversi

sulla consistenza dei residui e sulle autorizzazioni definitive di cassa, ricollegabili a discordanze relative ai pagamenti disposti mediante ruoli di spesa fissa, nonché a pagamenti di titoli del debito pubblico, nonché le spese effettuate in mancanza di stanziamenti in bilancio, registrate nel consuntivo come eccedenze, verificatesi in capitoli dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'istruzione dell'università e della ricerca, delle infrastrutture. Nel dettaglio, la Corte dei conti ha rilevato la presenza di discrasie in ordine all'esistenza di eccedenze di spesa sulle previsioni definitive di competenza, sulla consistenza dei residui e sulle autorizzazioni definitive di cassa. Anche per il 2012 non è mancata una serie di capitoli di cui non è stata prodotta la certificazione delle risultanze finali del conto dei residui, in quanto al momento dell'approvazione del referto non sono stati approvati dalla Corte dei conti i relativi decreti di accertamento. Sulla questione dei residui attivi e dei residui passivi, la Corte continua ad insistere. Alla base della perdurante anomalia del fenomeno dei residui passivi, pur sottolineando miglioramenti rispetto all'anno precedente, si collocano molteplici e diversificate cause: le misure di contenimento della spesa non sempre rispettate, spesso orientate allo slittamento dei pagamenti; la cattiva qualità della legislazione, non sempre supportata da specifici progetti di fattibilità; le procedure complesse e defatiganti in alcuni settori di intervento, gli schemi contabili spesso obsoleti; gli incongrui comportamenti gestionali. Per quanto riguarda i residui attivi, la Corte evidenzia le discordanze fra i dati del rendiconto e le contabilità di entrata delle amministrazioni e incongruenze interne al consuntivo. Anomalie, quelle relative ai residui attivi e passivi, che nel complesso mettono in crisi l'annualità del bilancio e la stessa rappresentatività del rendiconto. Sul punto si ribadisce l'esigenza di procedere ad un netto miglioramento delle metodologie di rilevazione contabile dei residui in misura tale da evitare qualsiasi ipotesi di aggiustamento fittizio dei conti pubblici. È noto, infatti, che l'andamento anomalo dei residui attivi e passivi potrebbe dare luogo ad un significativo *surplus* derivante dall'andamento differenziato dei medesimi che rischia di (o potrebbe) contribuire in misura non irrilevante al miglioramento dei saldi. La Corte dei conti solleva preoccupazioni anche in merito alla trasparenza del bilancio pubblico, sulla quale incidono alcune modalità di contabilizzazione delle voci. In tal senso, ad esempio, la Corte ha rilevato l'esistenza di resti da riscuotere delle entrate extratributarie classificate come di riscossione certa, quantunque ritardata, pari al 100 per cento, nonostante l'esiguo grado di realizzo, nonché 1'esistenza di poste di bilancio per le quali si sono rilevate minori entrate rispetto alle previsioni iniziali e definitive di bilancio. La legge n. 196 del 2009 rende possibile ridurre l'impatto di tali criticità. La maggiore trasparenza ed analiticità delle risultanze di bilancio dovrebbe, infatti, consentire la verifica della correttezza della gestione e l'effettivo rispetto delle autorizzazioni disposte con il bilancio di previsione. È auspicabile a tal fine che già a partire dal prossimo anno il rendiconto divenga un valido strumento conoscitivo e di supporto alle valutazioni del Parlamento e della Corte dei conti circa l'allocazione a consuntivo delle risorse tra le funzioni assolte dall'intervento pubblico e l'effettivo conseguimento degli obiettivi assegnati a ciascuna amministrazione. Perché questo si verifichi è tuttavia necessario un deciso rafforzamento dell'azione di controllo svolta dal Parlamento e, innanzitutto, dalle Commissioni permanenti. Occorrerà, infatti, sviluppare la capacità di monitorare in profondità l'attuazione finanziaria delle missioni e dei programmi coinvolgendo i responsabili della spesa dei singoli Ministeri. Tale attività non potrà essere limitata alle Commissioni bilancio e dovrebbe giovarsi dell'esercizio della delega prevista dall'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, relativa alla revisione della struttura del bilancio, che dovrà intervenire su un'articolazione delle missioni e dei programmi per molti aspetti inadeguata e scarsamente rappresentativa delle effettive linee delle azioni di amministrazione. Questo è il nostro auspicio. In conclusione, considerata l'importanza che riveste il rendiconto 2012 anche in relazione alla prossima sessione di bilancio, si auspica l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

Presidente, colleghi, membri del Governo, il disegno di legge di assestamento per il 2013 evidenzia anzitutto un peggioramento dei saldi di bilancio in termini di competenza rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2013. Il saldo netto da finanziare passa infatti da - 6.185 milioni a - 31.065 milioni, con un peggioramento di 24.881 milioni, pari a circa il 400 per cento rispetto all'entità del medesimo aggregato indicata dalla legge di bilancio; detto importo deriva dalla somma di un peggioramento di 15.029 milioni, dovuto a variazioni per atto amministrativo, imputabili prevalentemente all'incremento delle spese per 16.586 milioni. In particolare, vanno ricordati l'avvenuta istituzione, disposta dal decreto-legge n. 35 del 2013, del fondo finalizzato ad assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, ed un peggioramento per 9.851 milioni derivante dalle proposte dell'assestamento stesso, riconducibili alle minori entrate finali, per un importo pari a 12.356 milioni, risultante da una forte diminuzione delle entrate tributarie (per 14.521 milioni) solo in parte compensata dall'aumento delle entrate extratributarie (per 2.088 milioni) e dalla vendita ed ammortamento di beni patrimoniali, pari a 77 milioni. Nell'ambito delle entrate tributarie, voglio sottolineare la contrazione del gettito IVA, per 10.548 milioni, nonostante l'aumento di un punto percentuale dal 20 al 21 per cento, di quello riveniente dall'accisa sui prodotti energetici, per un importo di 4.257 milioni, dal bollo, per 2.011 milioni, mentre, al contrario, le previsioni dell'IRPEF, dell'IRES e dell'imposta sostitutiva registrano un aumento pari rispettivamente a 2.803 milioni, 1.599 milioni In merito al predetto andamento delle entrate, avevo rilevato in Commissione bilancio come il gettito IRPEF risulti generalmente correlato positivamente con il livello dell'occupazione e del PIL, il gettito IRES con il PIL, e il gettito IVA con la dinamica dei consumi e delle spese delle famiglie, nonché con le importazioni, chiedendo pertanto aggiornamenti degli indicatori economici al Governo, atteso che le principali componenti della domanda interna sono previste in forte contrazione rispetto al 2012. Il Governo ha riferito in proposito che, sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito nei primi sette mesi dell'anno, nel complesso le le entrate tributarie contabilizzate al bilancio dello Stato, proiettate su base annua, risultano sostanzialmente in linea con quelle contenute nel bilancio di assestamento, sulla base di alcune considerazioni che sintetizzo. In primo luogo, il gettito dei primi sette mesi del 2013 è atteso crescere dell'1,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ovvero ad un tasso superiore al tasso di crescita delle entrate tributarie assestate per il 2013 rispetto al consuntivo 2012. Il gettito IRPEF, anche se correlato al PIL e all'occupazione, mostra a tutto luglio una crescita dell'1,1 per cento, ascrivibile essenzialmente agli incrementi delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico dovuto agli effetti dei conguagli fiscali e dei versamenti in autoliquidazione. Tali incrementi compensano ampiamente la lieve flessione delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato (-0,5 per cento) e quella più marcata sui redditi dei lavoratori autonomi (-6,0 Per quanto concerne l'IRES, essa ha mostrato al contrario una crescita assai significativa nel 2013 rispetto all'anno precedente, pari al 12,8 per cento, soprattutto per effetto di consistenti versamenti IRES effettuati da parte di grandi contribuenti del settore bancario e assicurativo. altre imposte dirette, contribuiscono al buon andamento delle entrate l'incremento acquisito nei primi sette mesi dell'anno delle varie imposte sostitutive. Infine, per quanto concerne il gettito dell'IVA,

ascrivibili per la gran parte alla spesa in conto capitale. La spesa corrente cresce, invece, in misura lieve (0,24 per cento, pari a 954 milioni) al netto degli interessi. Per i benefici dell'inventario, ritengo utile ricordare che a fine anno la spesa per interessi sul debito dello Stato sarà pari a 89.162 milioni (500 milioni in meno rispetto alle previsioni). Passando all'assestamento delle previsioni in termini di cassa, si rileva che anche queste determinano, nel 2013, un peggioramento dei saldi. Il peggioramento del saldo netto da finanziare è di 29.187 milioni di euro (si passa cioè dai 73.691 milioni delle previsioni iniziali a 102.878 quello del risparmio pubblico di 15.512 milioni (si passa da 28.075 a 43.587 milioni). Il saldo primario peggiora

mentre il ricorso al mercato, infine, peggiora di 24.546 milioni (da 284.489 milioni a 309.035 milioni). Tralascio per ragioni di tempo le considerazioni

interventi normativi effettuati con i decreti-legge nn. 98 del 2011, 138 del 2011 e 95 del 2012. quindi ad illustrare l'articolo 2 del provvedimento in esame. Va anzitutto rilevato che esso contiene alcune modifiche rispetto alla legge di bilancio per il 2013. In particolare, il comma 1 dispone l'aumento dell'importo autorizzato di emissione dei titoli pubblici, portandolo portandolo da 24 (come stabilito dall'articolo 2, comma 3, della citata legge di bilancio) a 80 miliardi di euro. A tale proposito, il Governo ha fatto presente che tale incremento delle emissioni nette miliardi è necessario per assicurare la liquidità necessaria alla copertura del maggior fabbisogno dello Stato, legato al pagamento dei 20 miliardi conseguenti all'applicazione del decreto-legge n. 35 del 2013, che sarà oggetto di uno specifico emendamento che prevede addirittura un ulteriore incremento del limite delle emissioni nette a 98 miliardi. L'incremento proposto permetterà, inoltre, di compensare i possibili sfasamenti inframensili fra incassi e pagamenti e di affrontare i primi mesi del 2014 con una sufficiente riserva di liquidità, senza mettere sotto pressione le emissioni all'inizio dell'anno, anche in considerazione della prevista accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali della pubblica amministrazione nella prima parte del 2014 (si prevede un incremento dei pagamenti dei debiti, anche quelli attuali, di Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che, al comma 7 dell'articolo 2 della legge di bilancio 2013, l'importo di 1.900 milioni è sostituito dall'importo di 2.000 milioni. L'incremento in oggetto riguarda il fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa. L'articolo 3 del provvedimento in esame aggiunge all'articolo 8 della legge di bilancio 2013 il comma 12-*bis* il quale, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, estende all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010 secondo il quale le suddette somme sono versate, a cura delle amministrazioni interessate, sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, istituito per ogni singola amministrazione. Signora Presidente, colleghi, onorevole Sottosegretario, in conclusione i dati contabili dell'assestamento evidenziano numerose criticità di gestione del bilancio. Si tratta, in primo luogo, del già accennato netto peggioramento dei saldi di bilancio in termini di competenza, con il saldo netto da finanziare che peggiora di circa il 400 per cento, anche a causa della contrazione del gettito IVA per oltre 10 miliardi Non ci possiamo nascondere che le manovre di correzione dei conti pubblici per il 2012 hanno sì consentito il miglioramento di alcuni saldi (peraltro solo di alcuni e in misura minore di quanto ci si sarebbe potuto attendere), ma hanno generato anche effetti depressivi sull'economia, come dimostra il calo delle entrate tributarie già in difficoltà e in forte recessione. Le cifre dei dati di bilancio fanno intravedere una situazione socioeconomica molto preoccupante: la disoccupazione in aumento, l'impoverimento di sempre più estesi strati di popolazione, la chiusura di piccole e medie imprese, la mancanza di sviluppo. Né le prospettive future appaiono migliori ove si consideri che, secondo le previsioni più aggiornate, riportate nelle considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia all'assemblea dei soci del 31 maggio 2013, anche quest'anno si chiuderà con un forte calo dell'attività produttiva e dell'occupazione. A questi andamenti si aggiunge quello ancora più preoccupante costituito dall'andamento del debito pubblico, che ha ampiamente superato la soglia di 2.050 miliardi di euro e si avvicina ai 2.100 miliardi altro che pareggio di bilancio previsto in Costituzione! Il Governo, inoltre, come accennato, si prepara a proporre un emendamento che incrementa l'importo massimo autorizzato di emissione dei titoli pubblici, portandolo da 24 a 98 miliardi Sin dal suo insediamento il Governo aveva promesso l'avvio di un'incisiva azione di *spending review* ma, ad oggi, a parte la norma che prevede di nominare un commissario *ad hoc*, ancora non abbiamo riscontrato effetti. si susseguono provvedimenti di maggiore spesa coperti da ipotetiche maggiori entrate: l'ultimo esempio è il decreto-legge n.91, il cosiddetto decreto valore-cultura, che all'articolo 14 incrementa la misura delle accise sugli oli e sull'alcol. Ulteriori spese si preannunciano nel decreto-legge in tema di pubblica istruzione approvato ieri dal Governo e ulteriori spese sono contenute nel decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione sulle pubbliche amministrazioni, con sanatorie di 100.000-150.000 precari. Si tratta, colleghi, di una gestione della finanza pubblica sulla quale non si può non nutrire riserve sia come cittadini che come operatori economici e come responsabili politici. Serve una riflessione e, se non basta, è necessario auspicare un cambio di rotta.

richiesto. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta. È iscritto a parlare il senatore Lai. Ne ha facoltà. *(PD)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, il provvedimento di assestamento del bilancio pubblico, oggi all'attenzione di quest'Aula è un passaggio importante del ciclo di bilancio con il quale si esamina lo stato delle nostre finanze pubbliche in corso di anno rispetto alle previsioni del bilancio approvato lo scorso dicembre 2012; un provvedimento che assume i dati relativi alle entrate e alle spese del primo semestre per adeguare il bilancio preventivo. Questa circostanza giunge a proposito per ricordare a tutti noi e, per nostro tramite (con l'aiuto dei *media)*, ai cittadini italiani che l'Italia non ha un'economia in equilibrio: non ha risolto tutti i suoi problemi non ha soprattutto le spalle sufficientemente larghe per sopportare qualunque carico, anche se *partner* importanti della maggioranza hanno previsto tali carichi nel loro programma elettorale. L'Italia può ripartire. Questo Governo ha intrapreso la strada opportuna, ma il percorso nasconde ostacoli dietro ogni angolo, soprattutto se non operiamo in un contesto di verità e se non siamo onesti con noi stessi. infatti, vent'anni di verità parziali o di vere e proprie bugie che ci hanno portato a questo punto e non un destino cinico e baro. Sono stati lunghi anni di impegni che non si potevano mantenere né si dovevano prendere, anni di scelte di Governo spesso lontane da ragionevoli valutazioni sullo stato di salute e sulle prospettive di crescita del Paese. Sono queste scelte che hanno portato il tasso di disoccupazione giovanile

Sud. Il provvedimento in esame, pur evidenziando dati nettamente migliori rispetto a quelli dello scorso anno e degli anni precedenti, ci ricorda dunque che il Paese non è in grado di garantire il mantenimento di promesse impossibili: lo confermano i 10 miliardi di euro in meno sull'IVA, i 4 miliardi di euro in meno sulle accise e anche i 2 miliardi di euro in meno sui questo anno: contrazioni che valgono quanto una manovra. Lo dimostra anche il *trend* dello *spread*, che in queste ore vede il recupero della Spagna sull'Italia dopo quasi due anni. lato ci danno coraggio i dati sul rallentamento della contrazione del PIL e la possibilità che alla riduzione di questa caduta possa corrispondere, il prossimo anno, un primo rimbalzo e una ripresa della crescita, ma sbaglieremmo a pensare che con la ripresa e la nostra capacità di agganciarla la nostra fiducia la credibilità internazionale siano raggiunte ed acquisite una volta per tutte. Per questo motivo il nostro Paese non può permettersi politiche da promesse elettorali, né di disperdere il patrimonio di credibilità di questi ultimi due anni che ha portato all'uscita dalla procedura di infrazione. Un obiettivo che al mio partito è costato in termini di consenso ma i cui risultati ci stanno consentendo le prime politiche espansive sostenibili da molti anni a questa parte. In questi due anni, a partire dalla fine del 2011, abbiamo chiesto ai cittadini e alle imprese italiane di sopportare manovre mai viste prima; l'intero Paese ha dovuto affrontare sacrifici enormi per mantenere gli impegni presi dal Governo precedente per il raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio. Spesso abbiamo anche discusso in merito agli impegni presi, chiedendoci se fossero eccessivamente gravosi, con il paradosso che spesso chi più li criticava era anche parte del Governo che li aveva assunti. Noi intendiamo confermare un giudizio positivo sul risultato ottenuto, dando merito però a chi più ha sacrificato per ottenerlo: imprese e cittadini. È il lavoro svolto in quei mesi che ha portato alla previsione di un rapporto *deficit*-PIL del 2,4 per cento per il 2013 e all'uscita dalla procedura di infrazione. Dopo molti anni si sono così aperte prospettive concrete e sostenibili di politiche espansive. La prima scelta di questo Governo è stata quella di confermare come impegni alcune scelte che erano state ipotizzate per favorire il rilancio economico già prima delle elezioni politiche di febbraio.

e per dimensione, fra le politiche espansive: ricordo quella per il mantenimento degli ecobonus ed i provvedimenti sull'occupazione sia quelli per i giovani, che quelli di salvaguardia del tessuto sociale ed imprenditoriale consentite dal rifinanziamento della cassa integrazione in deroga.

Tutti questi provvedimenti sono stati resi possibili grazie a politiche finanziarie rigorose quanto rispettose dei parametri condivisi in sede europea. Ora ci troviamo ad un bivio. Non si tratta tanto di scegliere tra stabilità o instabilità perché politiche inadeguate, per quanto in un contesto di stabilità, non produrranno la capacità del Paese di agganciare la ripresa; si tratta invece di scegliere se confermare il percorso che ci ha consentito di rientrare nei parametri e di considerare quello come il faro indispensabile che consente politiche espansive, oppure pensare che il risanamento sia acquisito una volta per tutte per tutte e torni ad una stagione di promesse facili con coperture finanziarie creative quanto improbabili. L'esempio nostro quanto quello di altri Paesi dimostra che queste politiche sono come le bugie, hanno le gambe corte, e per questo fanno fare poca strada. Lo dico perché c'è chi pensa di alzare continuamente l'asticella al Governo, ritenendo che le politiche economiche dell'esecutivo Letta possano essere quelle del programma elettorale di uno o dell'altro partito, sommando le necessità e le promesse piuttosto che facendo scelte. scelte. Su questo fronte il Paese non può permettersi di andare indietro; la stabilità non è raggiunta una volta per sempre e il rischio di vanificare gli sforzi fatti dagli italiani nel 2011 e nel 2012 è presentissimo.

Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi senatori, affermava Schumpeter all'inizio del Novecento, che il bilancio dello Stato è lo specchio di tutti i problemi politici e sociali di una Nazione. le tabelle poco attraenti del bilancio che si esplica la politica economica che lo Stato persegue; dal bilancio ricaviamo quali sono le politiche di stabilizzazione, di crescita, di redistribuzione e riallocazione delle risorse. Il rendiconto e l'assestamento sono un prolungamento del bilancio; permettono la gestione dinamica dello stesso in seguito a mutamenti dello scenario economico e di nuovi atti normativi. In questa ottica, il dibattito su rendiconto e assestamento dovrebbe essere rivitalizzato, dovrebbe uscire dalla cerchia ristretta degli esperti e diventare dibattito pubblico, aperto a tutti i cittadini. Questo migliorerebbe certamente le relazioni tra la politica e la cittadinanza. Ancora oggi, invece, il rendiconto e l'assestamento sono di difficile comprensione e il loro linguaggio è spesso ostico. Benché l'obiettivo del rendiconto sia quello di valutare se la gestione dell'esercizio concluso al 31 dicembre sia stata finanziariamente corretta, se gli obiettivi siano stati conseguiti e le risorse finalizzate allo scopo siano state sufficienti, una lettura dell'Atto Senato n. 888 non permette facilmente tali valutazioni: ad esempio, non è possibile sapere quali siano stati gli effetti della *spending review*, quale l'efficacia delle politiche per i Ministeri,

del Senato e della Camera in merito agli atti di indirizzo che assumiamo. Inoltre, l'articolo 36 della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) stabilisce che il rendiconto generale dello Stato è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. Eppure, dal rendiconto presentato, questo secondo aspetto legato al patrimonio non è sufficientemente chiaro: dal rendiconto non è possibile sapere quale sia la valutazione del patrimonio dello Stato, nonostante uno degli obiettivi della nuova legge di contabilità (la citata legge n. 196 del 2009) sia stato proprio quello di semplificare il bilancio e rendere più chiara la comunicazione verso i cittadini.

un elemento strategico, se vogliamo anche moralizzare i nostri stessi conti. Metterò ora rapidamente in evidenza alcune questioni legate ai disegni di legge in oggetto,

all'andamento negativo dei proventi legati ai giochi. Rispetto alla prima questione, sottolineo che la forte flessione del gettito dell'IVA, così come di altre imposte sui consumi, deriva dal fatto che nel 2013 la riduzione del livello dei consumi interni ha raggiunto la sua fase più acuta; anche oggi abbiamo avuto ulteriori attestazioni della situazione di grave problematicità a tale riguardo. Viceversa, si è registrato un andamento positivo per le esportazioni. Un ulteriore fattore che ha inciso sulle entrate IVA è stato anche il ritardato versamento dell'imposta da parte delle aziende colpite da una crisi di liquidità. A questo proposito è importante sottolineare che il Governo, come assicurato in Commissione, proceda a un attento studio sulla misurazione dell'impatto macroeconomico sui consumi di misure di aumento del prelievo IVA, anche per valutare la relazione sussistente tra consumi, aspettative dei consumatori e incremento di aliquota. Così come è importante che al più presto si proceda al totale pagamento dei debiti arretrati della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese affinché quel problema di liquidità che si riscontra - ahinoi! - nella voce «mancate entrate» possa in qualche modo ridursi. Per quanto riguarda la flessione delle entrate nel settore dei giochi, sembra che essa derivi da un aumento dei livelli di povertà, tenendo presente che una maggiore propensione al gioco si registra proprio nell'ambito delle categorie con reddito medio-basso. Anche in base al dibattito svoltosi la scorsa settimana al Senato sugli effetti dell'azzardo (più che del gioco, come è stato ricordato), è importante che il Governo si impegni sul fronte del contrasto al gioco lecito ed illecito,

Ancora qualche breve osservazione sul rendiconto. Le previsioni definitive delle spese sono aumentate rispetto a quelle iniziali del 3 per cento. L'aumento ha riguardato le categorie: trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, consumi intermedi, trasferimenti correnti alle imprese e redditi da lavoro dipendente. L'incremento delle previsioni per spese in conto capitale è da ricondurre principalmente alla sottoscrizione al capitale del meccanismo europeo di stabilità. Per quanto riguarda i saldi, il risparmio pubblico, vale a dire il saldo tra le entrate correnti, tributarie ed extratributarie, e le spese correnti, ha evidenziato un miglioramento. Questo è certamente un dato importante da sottolineare. Rispetto all'esercizio passato c'è un evidente cambio di tendenza, passando da un valore negativo di 606 milioni di euro in perdita al valore positivo registrato nel 2012 per cento). Tuttavia le variazioni proposte con l'assestamento fanno registrare una previsione di 24.346 milioni, in peggioramento rispetto alle previsioni del bilancio 2013. Ancora una volta la crisi si

Anche l'avanzo primario è superiore di 17.505 milioni rispetto a quello del 2011. Guardando i dati del rendiconto economico delle amministrazioni, dall'esame dei dati emerge il peso degli interessi sul debito debito (è l'ultimo dato che vi fornisco), pari al 18 per cento del totale generale, che è di poco inferiore ai costi propri (personale, beni e servizi) di tutte le amministrazioni centrali, a loro volta pari al 20 per cento del totale generale.

innanzitutto sottolineare, come già fatto dal primo collega intervenuto in discussione generale, che la legge di approvazione del rendiconto rappresenta una formale approvazione da parte di questo Parlamento degli atti di gestione realizzati nell'anno finanziario. Non si tratta, dunque, di un mero atto simbolico: si tratta di una presa di coscienza, di un'approvazione molto importante. È bene quindi che prima di analizzare questi atti ed esprimere un voto si faccia un'attenta riflessione su quello che questi atti rappresentano. Per quanto riguarda il MIUR, dunque, a prima vista nulla di scandaloso quando si legge nel rendiconto del 2012 che gli stanziamenti di competenza ammontano a 53,1 miliardi di euro e 54,2 miliardi di euro sono le autorizzazioni di spesa. Questo risultato però è pervenuto - lo ricordo - dopo gli anni di contenimento della spesa, che hanno avuto origine nel famigerato articolo 64 della legge Gelmini. È molto interessante segnalare a questa Assemblea, a voi tutti, alcune considerazioni che a tal proposito fa la Corte dei conti, e che sono presenti nella relazione che la Corte ha presentato unitamente ai disegni in questa relazione si legge che l'analisi finanziaria del bilancio del MIUR ha evidenziato, sul fronte delle spese, una consistente riduzione delle risorse assegnate.

la riduzione dei servizi a tutti, in particolare ai disabili e agli studenti di origine straniera, il ridimensionamento degli orari, di discipline, di sperimentazioni nelle scuole superiori, la carenza di fondi per l'ordinario funzionamento delle scuole per qualsiasi progetto didattico. I tagli cui si fa cenno per il triennio 2009‑2011 sono di ben 7,8 miliardi di euro e 130.000 posti sono stati persi negli organici del personale della scuola; solo per il personale ATA i tagli costituiscono il 35 per cento dell'organico tra il 2008 e il 2013, e merita attenzione anche segnalare che tutto questo è avvenuto mentre gli studenti aumentano. Nel primo anno di tagli (anno scolastico 2009‑2010) gli alunni sono aumentati di 40.000 unità, ma sono stati assegnati

Questa non completa realizzazione è ascrivibile, in particolare, al ritardo nella riorganizzazione della rete scolastica, conseguente a due sentenze della stessa Corte costituzionale, la n. 200 del 2009 e la n. 147 del 2012,

conferma la validità delle misure di razionalizzazione poste in essere in attuazione del» - famigerato, dico io - «articolo 64 della legge n. Ma signori, secondo voi queste sono parole degne di un Paese civile? Stiamo dicendo che abbiamo sfasciato la scuola ma che non si è fatto abbastanza; ci si lagna di sentenze della Corte costituzionale che hanno cercato di dimostrare (e hanno dimostrato, perché i relativi ricorsi

che lo Stato, con regolamenti governativi, provvede alla definizione del ridimensionamento della rete scolastica, nonché a particolari misure nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici. Ebbene, questa previsione è anticostituzionale, perché va contro l'articolo 117 della Costituzione. L'altra sentenza della Corte costituzionale che costituisce una difficoltà è la n. 147 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità di un altro articolo di una legge del ministro Gelmini che prevedeva l'accorpamento della scuola dell'infanzia e della scuola primaria nella scuola secondaria di primo grado, aggregate in istituti comprensivi costituiti di almeno 1.000 alunni. Anche questa previsione è incostituzionale. Anche questo è stato fatto. La Corte costituzionale, accogliendo tutte queste motivazioni dei ricorsi presentati dalle Regioni, stabilisce una chiara linea di demarcazione tra le competenze dello Stato È opportuno quindi sottolineare che queste difficoltà, contrassegnate dalla Corte dei conti non sono semplicemente dovute a ritardi, ma al fatto che i provvedimenti contenuti nella legge Gelmini sono illegittimi e incostituzionali. *(Applausi Per non parlare della sentenza n. 80 del 2010, in materia di posti di sostegno, che è ancora più grave, perché ribalta la situazione, del tutto inopportuna e allucinante, che si era venuta a creare a seguito della riforma Gelmini, in cui le risorse per il sostegno venivano decise a livello centrale e poi distribuite alle Regioni senza tenere conto delle specifiche esigenze degli alunni diversamente abili.

Ebbene, noi, come Movimento 5 Stelle, lo esamineremo con spirito costruttivo, come abbiamo sempre fatto; vorrei però sottolineare che il modello di scuola che esce da questo rendiconto dello Stato 2012 e dall'assestamento 2013 non solo ha mortificato la dignità degli alunni, degli insegnanti e del personale ATA, che lavorano con dedizione, assicurando un livello che non sarebbe possibile con le risorse assegnate,

l'occasione del dibattito sul conto consuntivo 2012 e sull'assestamento 2013 è per tutti noi una fondamentale tappa per revisionare in maniera critica il motore stesso della nostra economia la rotta che stiamo dando al percorso di risanamento e rilancio, per verificare la bontà e l'incisività delle nostre scelte strategiche, come pure per orientare perfino le nostre valutazioni sui Governi, la loro qualità e la loro durata. Forse, e lo dico con profondo rammarico, questo mio *incipit* è totalmente smentito dalle cronache di questi giorni che poco o nulla riportano di quanto qui stiamo effettivamente compiendo. È il rito stanco, stantio, del nostro Paese: l'abitudine di non addentrarsi nella concretezza delle scelte e soprattutto nella loro quantificazione economica, lasciando che questa divenga materia di pochi nella quotidianità che decide, e di tutti nei commenti che stroncano superficialmente. Probabilmente a questo concorre anche «osticità» con cui noi trattiamo la materia, come sottolineava molto bene poco fa il collega Olivero. Eppure avremmo veramente tanti e validi motivi per fermarci, anche per settimane, a lavorare su questi numeri. Il 2012 è stato un anno cruciale, per certi versi orribile, per certi altri ancora di svolta. Costretti a dover scegliere tra austerità e crescita, almeno nell'immediato, tra il timore di trascinare, con ristrettezze ulteriori, la crisi dentro un vortice depressivo e la consapevolezza che le mancate riforme del passato rendevano, come rendono ancora, la macchina pubblica praticamente inservibile allo scopo di fungere da traino, in un momento in cui ce ne sarebbe stato Sono queste le scelte sofferte che vanno conosciute e rintracciate dentro il consuntivo e sempre questo è il segno e la tendenza che occorre valutare criticamente nel comporre l'assestamento per il 2013. È di questi giorni, delle ultime settimane, la previsione sempre più insistente e confermata di un rallentamento della crisi anche per il nostro Paese e di un ritorno ad un terreno positivo, almeno per i consumi. Eppure abbiamo pagato e stiamo pagando un prezzo altissimo più degli altri grandi Paesi europei. In ciò, dentro questo ritardo, questa pesantezza, questa deriva, forte è il peso negativo della nostra macchina pubblica che, più di ogni altro sistema europeo, aggrava una già fiaccata economia reale con una tassazione che ha passato forse ogni livello di guardia, senza fornire, attraverso la spesa pubblica, servizi che siano equiparabili alle dimensioni di questo sacrificio. Anche il 2012 ci ha visti dentro questa morsa, la morsa di una pressione fiscale ancora impossibile da calare, anzi in aumento, e di una spesa pubblica non intaccata dalla revisione di cui abbiamo bisogno. A nessuno sfugge che questo pericoloso stallo, che riguarda il bilancio pubblico con evidenti e pesanti riflessi e condizionamenti sul settore privato, è reso particolarmente bloccato e statico dalla mole del debito e degli interessi sul debito, che praticamente vanificano la virtuosità di un avanzo primario positivo, che anche lo scorso hanno è stato Vanno però riconosciuti, con il rammarico fin qui espresso sulla mancata corrispondenza in termini di incisività rispetto a quanto il Paese avrebbe necessitato, gli inequivocabili segnali di buona tendenza, quali, ad esempio, il miglioramento del saldo sulla spesa di parte corrente, che nel 2012 ha continuato ad essere negativo, ma di «soli» 6 miliardi di euro, a fronte degli oltre 23 miliardi dell'esercizio precedente. Accanto a questo dato positivo, dobbiamo tuttavia registrare il crollo degli investimenti per quanto riguarda il nostro Paese. Questo sforzo viene peraltro immediatamente compensato, in negativo, dal dato sugli interessi passivi (ricordiamo tutti le vere e proprie sofferenze legate all'andamento dello *spread* BTP-BUND), che registrano un incremento anno su anno del 10,4 Si rifletta attentamente su questo aspetto, su quanto possa incidere ed incida, nei nostri conti pubblici, la credibilità e la solvibilità del sistema, costituendo di fatto una tassa, tutt'altro che occulta e del tutto improduttiva. Pensando agli sforzi compiuti ad ogni livello dello Stato, che vengono piuttosto brutalizzati dentro ai numeri di questo consuntivo, si possono rintracciare elementi di soddisfazione per aver neutralizzato possibili effetti negativi e distruttivi di una tempesta finanziaria che ci ha investiti. Devono anche sorgere, però, nuove preoccupazioni che inducano a mettere mano, con maggior vigore e sistematicità, alla revisione della spesa e all'abbattimento del debito, due lame che pericolosamente si avvicinano come una forbice posta sul nostro futuro. Questo consuntivo, forse sincopato rispetto ai nostri bisogni, privo di elementi che facciano emergere entusiasmi sia per chi voglia auspicare una mano pubblica generosa negli investimenti, che per chi ne richieda un alleggerimento nei prelievi, ha dentro di sé il valore di un'inversione di tendenza, o meglio, di una continua inversione di tendenza, considerati anche gli anni immediatamente precedenti, con l'innegabile pregio di averci portato all'uscita dalla procedura di infrazione e di aver aperto quegli spazi che ci hanno consentito di liberare risorse (penso allo sblocca-crediti e agli altri interventi ricordati poco fa), in un momento che si è rivelato cruciale per impedire una caduta verticale e consentire di guardare al finale dell'anno con maggiore serenità. Possiamo ben dire, e ne siamo convinti, di avere evitato il peggio, di avere messo in sicurezza i conti pubblici. Ma siamo solo al principio della nostra opera: a nulla vale questa virtuosità finché non si rifletterà in miglioramento effettivo per i nostri cittadini. Non commettiamo nuovamente gli errori del passato. Non distraiamoci e perseveriamo nell'opera di risanamento, di cambiamento e di rilancio dell'economia. Diamo vita ad azioni straordinarie che ci consentano di rompere le catene di cui ormai tutti tutti siamo consapevoli e mettiamo lo Stato e le nostre istituzioni nelle condizioni di concorrere all'intrapresa dei cittadini, di sostenerla e promuoverla come dovrebbe essere. Signora Presidente, continuiamo e rafforziamo quest'opera di risanamento e rilancio cui va la nostra approvazione. Signora Presidente, approfitto di questo breve intervento per riportare anche a questa Assemblea la riflessione che ho già condiviso con i colleghi della Commissione finanze riguardante il provvedimento di assestamento del bilancio. Leggiamo nella relazione introduttiva che una delle motivazioni che ha reso necessario tale assestamento è stato il minore gettito fiscale, con riferimento, in particolare, alle imposte indirette, giustificabile dalle evidenti criticità del quadro macroeconomico. Nell'ambito di queste ultime, un peso consistente ha la riduzione del gettito IVA, quantificato in circa 10 miliardi di euro. Il paradosso è già evidente: a fronte di un aumento dell'aliquota IVA di un punto percentuale, il gettito complessivo diminuisce, logica conseguenza di un mercato interno in forte sofferenza, situazione che trova purtroppo conferma anche nei dati congiunturali dei primi mesi del 2013. Nel corso della seduta di Commissione, il vice ministro Casero ci ha informato del fatto che si sta studiando la correlazione tra aumento dell'imposta e diminuzione della domanda interna, precisando, tuttavia, che al variare del quadro economico complessivo, in uno qualsiasi dei suoi elementi, non è detto che tale correlazione rimanga immutata. Tuttavia, valutando l'attuale situazione, non emergono elementi che facciano pensare ad una ripresa immediata della domanda interna, mentre alle porte si prospetta un nuovo aumento dell'aliquota ordinaria IVA. Sarà dunque banale, ma io non valuterei l'aspetto psicologico o il timore dei cittadini italiani per il futuro (che pure è evidente) che aumenta la propensione al risparmio, anche a fronte di un maggiore reddito disponibile. Piuttosto farei la semplice considerazione del consumatore: se costa di più ne compro di meno o magari non ne compro affatto. Si viene a creare una spirale perversa, per cui non solo ad ogni aumento dell'imposizione non corrisponde una maggiore disponibilità di fondi per l'erario, bensì una diminuzione degli stessi, ma anche una riduzione dei consumi, con conseguenze letali sul tessuto produttivo. A meno che, certo, qualcuno non pensi seriamente che questo possa mantenersi a tempo indeterminato sul solo *export*. Invito il Governo a leggere questa situazione come un ennesimo campanello d'allarme e ad effettuare una seria e profonda riflessione sull'opportunità e sull'utilità di aumentare ulteriormente l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto. Magari è vero che non c'è un legame diretto, magari è vero che è solo una questione psicologica, ma, alla luce delle notizie che quotidianamente ci riportano le mille difficoltà che molte famiglie italiane affrontano semplicemente per sopravvivere, davvero si è disposti ad aggiungere un'altra carta ad un castello già così traballante? Sotto il castello - ricordiamocelo sempre - ci sono i cittadini italiani e nel dubbio sarebbe bene non rischiare.

legge di assestamento è un atto importante perché, al di là dell'adempimento dell'articolo 33 della legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica, è l'occasione in corso d'anno di fare una verifica, non solo sui dovuti equilibri di bilancio, ma anche sull'avanzamento degli obiettivi che Governo e Parlamento vogliono conseguire nel corso del 2013. Il mio intervento riguarderà gli aspetti procedurali e temporali del i dati sull'assestamento e, in ultima istanza, la verifica del raggiungimento degli obiettivi. Poche battute sugli aspetti procedurali e temporali, non solo del nostro assestamento, ma anche degli altri atti che devono compiere gli enti locali. L'articolo 33 della legge di contabilità

Il rispetto dei tempi non è solo forma, ma è anche sostanza. Se occorre intervenire per modificare qualcosa, se non stiamo raggiungendo gli obiettivi, è bene non farlo alla fine dell'anno, ma a metà dell'anno, come giustamente prevede la normativa. Ma questa è un'abitudine tutta italiana: il decreto‑legge n. 102 del 31 agosto proroga al 30 novembre il termine per gli enti locali di approvare il bilancio di previsione per il 2013 e per l'approvazione del regolamento e delle tariffe della TARES. Come se non bastasse, sono rinviate ad ulteriori provvedimenti sia l'eliminazione dell'IMU (rata di dicembre), sia l'introduzione dal 2014 della *service tax*. Il metodo va in netta contraddizione con i principi della sana programmazione. Continuare con la gestione provvisoria fino al 30 novembre significa mettere a rischio gli equilibri di bilancio, soprattutto nella parte corrente. Ci vogliono ancora settimane per l'esatta quantificazione della copertura statale. Si può ancora chiamare bilancio di previsione un documento approvato con l'assestamento e che quindi non è più modificabile? Diventa sostanzialmente un preconsuntivo. È vero che il Governo ha vissuto con grande difficoltà questi mesi, ma auspico davvero che per il prossimo anno si possano rispettare i diritti delle autonomie e consentire loro di fare i bilanci nei tempi dovuti. Infine, sento di fare mio il suggerimento del Servizio del bilancio del Senato, che nel *dossier* n. 6 sostiene: «La Ragioneria generale dello Stato (RGS) comunica nella pagina *web* del proprio sito Internet dedicata a Open data che i dati relativi al lato spesa della legge di assestamento saranno rilasciati in formato elaborabile entro un mese dall'approvazione della legge stessa. A tale proposito, andrebbe valutata l'opportunità di provvedere ad una revisione di tale tempistica

poche osservazioni sui dati dell'assestamento. Rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, i dati contenuti nel disegno di legge, espressi in termini di competenza e considerati al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA, evidenziano un peggioramento dei saldi di bilancio. Il saldo netto da finanziare presenta una variazione di segno negativo di circa 25 miliardi, di cui 15 in relazione ad atti amministrativi e 10 derivanti dalle proposte dell'assestamento stesso. Ne risulta che, a fronte della previsione iniziale negativa della legge di bilancio 2013 (-6 miliardi), il saldo netto da finanziare, nelle previsioni assestate, presenta un valore negativo di 31 miliardi. L'incremento delle spese per atti amministrativi è da imputarsi in gran parte all'istituzione del fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti delle amministrazioni locali: quindi un dato negativo, ma che dobbiamo considerare come la giusta, corretta conseguenza di un provvedimento estremamente positivo per la nostra economia.

Al contrario, le previsioni dell'IRPEF, dell'IRES e dell'imposta sostitutiva registrano un aumento pari, rispettivamente, a 2,8, 1,6 e 1,2 miliardi. Per quanto riguarda l'andamento delle entrate, ricordiamo che il gettito IRPEF risulta in linea generale correlata positivamente con il livello dell'occupazione e del prodotto interno lordo, il gettito IRES con lo stesso PIL e il gettito IVA con la dinamica dei consumi e delle spese delle famiglie, nonché con le importazioni. Questo sta a significare alcuni segnali contraddittori. ricorda che «la legge di assestamento provvede generalmente a ridefinire il limite di emissione dei titoli per tener conto delle modifiche degli obiettivi di fabbisogno intervenute o previste nel corso dell'esercizio».

incrementato per consentire agli enti locali una maggiore possibilità di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Anche questo è un dato letto in senso negativo che va però a coprire un intervento estremamente positivo per la nostra economia. Infine, affronto l'ultimo aspetto. L'assestamento dovrebbe essere l'occasione per effettuare una verifica del raggiungimento degli obiettivi. La relazione al Parlamento presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze illustra alcuni impatti stimati sulle misure incluse nel decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, ed effettua un primo esame della situazione economica in vista dell'imminente presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2013,

I dati relativi al secondo trimestre 2013 ci dicono che il PIL è diminuito dello 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente e del 2,1 per cento rispetto al secondo trimestre del 2012, in peggioramento rispetto alle stime del 6 agosto. I principali aggregati della domanda interna (consumi finali nazionali e investimenti fissi lordi) sono diminuiti entrambi dello 0,3 per cento. Le esportazioni (unico dato positivo) sono aumentate dell'1,2

Tornando alla relazione del presidente Letta, si sostiene che il complesso delle nuove misure di agosto avrà un impatto favorevole sull'economia e lascerà inalterato l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, riflettendosi unicamente sul fabbisogno finanziario e sul debito. Le ultime informazioni disponibili sembrano confermare l'ipotesi avanzata dal DEF di una ripresa dell'attività economica nella seconda parte dell'anno. Già da alcuni mesi si sono manifestati si sono manifestati i primi segnali di una progressiva stabilizzazione del ciclo economico, ma il Presidente stesso evidenzia le criticità sulle previsioni di crescita annua contenute nel DEF che dovranno essere riviste verso il basso.

Il quadro non è roseo. L'instabilità ci punisce; la Spagna ci raggiunge sui livelli dello *spread* in questi giorni. Occorre dedicare tutte le nostre forze e il nostro impegno ad un'azione volta ad evitare la morte dei flebilissimi segnali positivi provenienti dall'economia e degli effetti positivi delle manovre che con tanta fatica abbiamo varato in questi mesi.

per sostenere una tesi. Badate, noi abbiamo iniziato questa legislatura prendendo atto dell'impossibilità di costituire un Governo omogeneo rispetto alle aspettative dello schieramento, per così dire, vincente, o meglio non perdente. Abbiamo indetto le elezioni primarie dove abbiamo messo in lizza candidati di primissimo ordine. C'è stato un travaglio che ha coinvolto tutti. Alla fine abbiamo fatto un Governo di emergenza per risolvere i problemi straordinari della nostra economia, sistemare la finanza pubblica, contenere il debito e consentire che il nostro sistema economico riprendesse a crescere e, quindi, risolvesse anche i problemi sociali, quelli della disoccupazione e della crescente povertà. Il risultato di questa vicenda, colleghi, è che oggi noi ci troviamo, alla vigilia quasi certa di con i conti riportati nel rendiconto dello Stato, ma anche e soprattutto nel provvedimento di assestamento del bilancio, che ci raccontano - non lo dico io, ma lo avete detto voi che siete i relatori di una situazione non preoccupante, ma allarmante, nella quale non torna giusto neppure uno dei conti che abbiamo fatto. Non abbiamo ridotto il debito

per agire sull'imposta indiretta esattamente come abbiamo agito sull'imposta diretta. L'IRPEF cresce con la disoccupazione che cresce. quindi spremendo quei pochi limoni che ancora hanno un pochino di succo fino a quando non ne avranno più. Questo è un Paese al declino; è disperato. È un Paese che rinuncia ad avere una prospettiva perché continua a macinare una risposta

Chiedete all'impresa: tollera questa risposta? No. Chiedete ai lavoratori: tollerano questa risposta? No. Nessuno la tollera. Allora perché l'abbiamo messa in campo e ci intestardiamo a sopportarla? Perché questa è l'indicazione degli organismi internazionali; questa è l'indicazione dell'Europa, cioè dei poteri politici ed economici più forti del nostro continente. Accettiamo così una condizione di subalternità, alla quale non c'è rimedio. Credo che noi non possiamo andare avanti così. Come hanno detto i relatori, è necessario un cambio di rotta. Allora, siccome adesso facciamo la fotografia e sappiamo che non stiamo funzionando bene, ma domani dobbiamo fare la legge di stabilità, qualcuno verrà con lo stesso tipo di proposta che ha avanzato fino ad oggi, a prescindere dal fatto che voi rimaniate insieme in questa maggioranza che non è anomala, ma è più di ogni altro aggettivo che sia reperibile nel vocabolario? Al di là del fatto che ci rimaniate voi o che venga qualcun altro a governare questo Paese, questo è il tipo di risposta che noi tutti possiamo reggere? Credo di no:

ragazzi, avete un microscopio che non finisce più. Ma noi non siamo in grado di reggere una situazione che misura la crescita con il microscopio. Abbiamo bisogno di un passo diverso.

Chiediamo misure organiche di politica economica che superino l'*austerity* a favore di interventi ed investimenti di sostegno alla domanda interna, sapendo selezionare,

sviluppo della nostra economia. Abbiamo detto più volte di partire dalle nostre vocazioni produttive e di non ammazzare la capacità di risposta delle situazioni locali. Abbiamo gestito questa fase con un progressivo accentramento, che non è solo nazionale, ma è anche europeo, e non funziona. Quelli che stanno in periferia non rispondono, perché non ci riconoscono. Noi chiediamo un piano per il lavoro. Ma le politiche del lavoro sono per forza politiche assistenziali, politiche passive, politiche che non rispondono ai bisogni di crescita del sistema economico, come d'altronde ho già detto. L'impresa nasce dal lavoro, dalla competenza, dall'applicazione delle persone. In questo modo è cresciuto il mondo. Bisogna prenderne atto. Chiediamo una diversa politica fiscale, più equa.

anziché uno perché la sua mobilità viene ridotta. Dobbiamo intervenire sull'assetto idrogeologico per non pagare i danni che si verificano in caso di pioggia. Risparmiamo sulla pulizia dei tombini delle città

Dobbiamo smettere di risparmiare stupidamente. Dobbiamo, cioè, utilizzare in modo migliore la leva del risparmio. Abbiamo bisogno di una politica industriale. Ma è possibile che abbiamo cinque milioni di cellulari nel Paese e non ne produciamo neanche uno? Di che cosa dovremmo vivere se rinunciamo ad avere una politica industriale, una politica di investimenti per la formazione, la conoscenza, la ricerca, la crescita

che abbiamo bisogno di modificare il prossimo assestamento di bilancio affinché preveda saldi diversi da quelli che abbiamo visto in questa circostanza.

e in prossimità di quello che da sempre è il provvedimento cardine per la programmazione economico-finanziaria del Paese, ovvero la legge di stabilità che a breve dovremo approvare, con il rendiconto e l'assestamento di bilancio si analizzano nel dettaglio voce per voce i capitoli che hanno determinato i risultati economici e finanziari dello Stato. Ebbene, cosa vediamo in tutti questi conti? conti? Numerosi e interessanti sono gli spunti di riflessione, tanto più che mai come oggi si rende necessario per un Paese come il nostro avere una fotografia della situazione economica quanto più analitica e approfondita. È noto infatti che il 2012 abbia rappresentato un anno di grandi, grandissimi sacrifici per i cittadini e per le imprese allorché su di essi sono gravati imposizioni fiscali e provvedimenti onerosi, primo fra tutti l'imposta municipale propria. Non è un caso del resto, come si può vedere sul rendiconto, che le entrate complessive tributarie sono sì aumentate rispetto alle previsioni fissate nel 2012, però non possiamo non sottolineare come si sia registrata anche una notevole diminuzione delle entrate relative alle imposte sul reddito, segno evidente di una difficoltà del sistema economico a creare nuova ricchezza e lavoro. Ad ulteriore riprova, nel 2012 il PIL nazionale si è assestato a 1.566 miliardi di euro, con una flessione in termini di volume pari al 2,4 per cento rispetto al 2011. È forse questo, onorevoli colleghi, il segno più evidente su cui ci dobbiamo concentrare; un segno di come le iniziative del Governo precedente non abbiano affatto portato quella crescita tanto decantata, ma anzi proprio come quegli stessi provvedimenti abbiano posto le basi per un'ulteriore recessione del sistema economico nazionale. Io mi ricordo che l'anno scorso, proprio in questo periodo, il professor Monti diceva era finita e che in fondo al *tunnel* c'era la luce. Ed io mi ricordo che gli risposi: ma è sicuro che non siano le luci del treno? Ci risulta difficile continuare a far credere agli italiani, quindi, che vi sarà una ripresa economica e che calerà il debito pubblico, quando lo scorso anno il famoso rapporto debito pubblico-PIL pubblico-PIL ha raggiunto l'incredibile valore *record* di 127 punti percentuali e oggi, invece, siamo arrivati quasi ai 130 punti percentuali. Resta il fatto, non a caso, che nel sistema fiscale italiano il problema non sia certamente rappresentato dal lato delle entrate, visto che almeno per quanto riguarda alcune Regioni d'Italia i cittadini lavorano alacremente pagando puntualmente quanto dovuto all'erario. Piuttosto, i problemi iniziano a manifestarsi quando si entra nello specifico del lato delle spese.

è di una chiarezza cristallina. Le previsioni definite delle spese complessive di competenza sono aumentate - ripeto, sono aumentate rispetto a una diminuzione dello 0,8 per cento manifestatasi nel precedente esercizio. in un momento di crisi, di grave crisi, in una fase nella quale tutti i cittadini stanno facendo sforzi enormi per riuscire a pagare le tasse tenendosi stretto un lavoro che per molti, purtroppo, è sempre più legato ad un filo, lo Stato, che dovrebbe dare l'esempio per una gestione corretta ed efficiente, cosa fa? Continua ad aumentare le sue uscite. Lo Stato, il primo attore di quella ripresa economica che noi tutti auspichiamo da tempo, è il primo che dovrebbe pianificare le iniziative per la ripresa e nei fatti è, invece, il primo che ostacola tale risalita. L'ennesimo paradosso dell'Italia, quindi, e nei fatti la cartina al tornasole perfetta di questo Paese. L'analisi del rendiconto però fornisce spunti notevoli anche per quel che riguarda le risultanze economiche dell'anno di ciascun Ministero, misurando con precisione i costi sostenuti dall'amministrazione centrale statale, suddividendo gli stessi tra costi di funzionamento e costi per trasferimenti di risorse finanziarie e pagamenti per interessi sul debito che lo Stato ha effettuato nell'anno.

derivanti dai tagli ai trasferimenti fornendo purtroppo così minori servizi ai loro cittadini, vi sono invece organi dell'amministrazione centrale dello Stato dove la terribile scure dei tagli pare non essersi abbattuta. Anzi (oltre al danno la beffa): la sensibile diminuzione registrata in questo capitolo deriva per lo più dai mancati reintegri del personale nella pubblica sicurezza, quando i recenti fatti di cronaca evidenziano quanto ci sia bisogno di maggior sicurezza

città! Insomma, stiamo continuando a tagliare sempre e solo ai soliti cittadini. Per questi motivi il Gruppo della Lega Nord nel corso

intento di tagliare i rami secchi e le inefficienze che costituiscono un pesante tappo per la ripresa del nostro Paese.

A tale proposito, la stessa Corte dei conti ha nuovamente censurato la pessima abitudine di spendere risorse senza prima averle adeguatamente coperte.

e aleatoria: ha utilizzato una copertura che non si sa se ci sarà. Solo attraverso una vera e concreta riduzione della spesa pubblica, il grande male di questa amministrazione (così come dimostrano chiaramente anche i due provvedimenti in esame) annunciare ai cittadini una vera ed efficiente riforma di uno Stato che, viceversa, rischia di continuare nel suo pericoloso avvitamento su se stesso.

sanno come spendere i soldi pubblici solo e soltanto per i propri cittadini. *(Vivi

cosa da dire: è il momento del coraggio! È il momento di fare un progetto chiaro ed efficace che guardi ai prossimi vent'anni da presentare agli italiani, chiedendo loro uno sforzo di unità su un'idea di futuro. Se ve la sentite e ce la sentiamo tutti insieme, lo possiamo fare. Naturalmente lo stesso progetto dovrà essere spendibile anche in Europa, facendo loro capire che è una strada possibile per uscire dalla difficile situazione nella quale siamo, senza nella quale siamo, senza incorrere in ulteriori infrazioni. È ovvio che non possiamo più agire sulla valuta per agire sulla nostra economia; è altrettanto chiaro che ormai la remunerazione del lavoro è talmente bassa che non permette di sopravvivere. Chi afferma il contrario, paragonandosi alla Cina, all'Est o all'India, dice una baggianata. Le infrastrutture e le politiche keynesiane non ci salveranno ed è finita l'era del cemento e degli enormi investimenti statali: quando fra quindici-venti anni quelle opere saranno pronte, risulteranno ormai obsolete e noi avremo pagato un prezzo altissimo, non solo dal punto di vista economico, ma anche ambientale. Ci rimane solo un fattore su cui fare leva: la qualità, in tutti i campi, anche la qualità della vita. Proprio per questo è il momento del coraggio.

Diamo un facile accesso al credito. Ripubblicizziamo la Cassa depositi e prestiti. Ridefiniamo i Trattati internazionali. Diamo supporto alle piccole casse rurali che potranno così facilitare e supportare la rete delle piccole e piccolissime imprese del loro territorio. Investiamo in cultura e formazione, sulla bellezza. Prendiamoci cura delle persone e dei luoghi nei quali vivono e lavorano. Disincentiviamo la grande distribuzione e i consorzi che si appropriano del 90 per cento dei finanziamenti. Semplifichiamo davvero la burocrazia. Attiviamo la lotta capillare a evasione, elusione e distrazione di fondi. Di CIPE e Infrastrutture SpA non parlo: mai mi sarebbe concesso abbastanza tempo. Come dicevo, è venuto il momento del coraggio: reinvestiamo l'avanzo primario per tre anni su un progetto chiaro ed efficace; facciamo una *spending review* degna di questo nome, con tagli mirati e coraggiosi e non più orizzontali, perché gli stessi tagli per tutti significano solo maggiori ingiustizie e mancanza di coraggio nelle scelte; abbandoniamo la difesa o almeno ridimensioniamola fortemente e investiamo su tutti i corpi che si impegnano per dare alla nostra quotidianità la serenità di cui tutti necessitiamo, con una particolare attenzione alla loro preparazione, al benessere e alle capacità degli uomini e delle donne che ci lavorano. Facciamo questo atto di coraggio, facciamo scelte diverse, invertiamo la rotta e portiamo l'Italia fuori da questo pantano. È iscritto a parlare il senatore Lai. Ne ha facoltà. signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi senatori, il Senato è chiamato ad approvare il rendiconto consuntivo per il 2012 e l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2013. Il dibattito sul rendiconto offre l'opportunità di una valutazione in ordine alla corrispondenza tra le previsioni di bilancio annuale e le risultanze della sua gestione. Si tratta di un momento, quindi, che permette al potere legislativo e a quest'Aula di verificare quella che è stata l'attività dell'Esecutivo durante l'esercizio precedente, naturalmente utilizzando il risultato di questa valutazione per correggere i conti dell'esercizio in corso. La discussione sui documenti di bilancio ci permette di operare, come di consueto in queste occasioni, alcune riflessioni sia di carattere specifico che di contesto più generale. *In primis* le cifre: i dati sul gettito tributario, esposti nell'assestamento 2013, in crescita nei primi sette mesi dell'anno in corso, ci inducono a riflettere. I risultati ottenuti dal fisco nei primi sette mesi dell'anno, come illustrati dal Governo in Commissione bilancio, hanno visto infatti il gettito crescere dell'1,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2012. Nel complesso, le entrate tributarie erariali registrate nel periodo gennaio-luglio 2013, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano infatti a 234.703 milioni di euro (più 2.770 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2012). Positivi anche i risultati ottenuti sul fronte delle entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo: 4.256 milioni di euro (più 287 milioni di euro pari ad un aumento del 7,2 per cento), a conferma, sottolinea una nota dell'Economia, «dell'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione». Sale dell'1,1% per cento il gettito IRPEF. In crescita anche il gettito derivante dalle imposte dirette, che registrano un aumento complessivo del 4,7 per cento (più 6.003 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il gettito IRPEF cresce dell'1,1 per cento (più 1.059 milioni di euro) trainato essenzialmente dagli incrementi delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico (più 3,8 per cento) e dei versamenti in autoliquidazione (più 2 Anche l'IRES presenta una crescita significativa del 12,8 per cento (più 1.965 milioni di euro), in particolare per effetto di consistenti versamenti effettuati da parte di grandi contribuenti. Il gettito IVA invece è in diminuzione. Sono segnali di sofferenza che giungono dal comparto della piccola e media impresa e dalle professioni. Sul piano della spesa, la decisione di parificazione del rendiconto da parte della Corte evidenzia quelle incongruenze contabili che il relatore al rendiconto ha già messo in evidenza e che non voglio ripetere. Su questo fronte occorrerà però potenziare lo strumentario conoscitivo del Parlamento in linea con quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge costituzionale n. 1

È la perdita di competitività della Lombardia, il motore economico d'Italia e una delle quattro regioni europee più forti economicamente (insieme al Rhône-Alpes, alla Catalogna e al Baden-Württemberg), a far retrocedere di posto il nostro Paese nella classifica UE delle regioni più competitive del continente. la Lombardia perde competitività penalizzata dalle disfunzioni del sistema Italia: dunque, un cane che si morde la coda. Risultato complessivo è che anche in Lombardia abbiamo assistito, negli ultimi anni, a un calo degli investimenti diretti esteri, indicatore questo assai eloquente dell'attrattività del territorio. Ebbene, da noi la quota degli investitori diretti esteri, già prima di tale brusco calo, era ancora molto lontana dallo *standard* europeo. Era pari cioè allo 0,8-0,9 per un terzo rispetto agli investimenti esteri in Francia, Germania e Regno Unito e un quinto rispetto agli investimenti fatti in Olanda. Tutto ciò si riverbera ovviamente sui dati macro- complessivi del Paese, dati che il relatore al rendiconto ha giustamente evidenziato. Gli ultimi dati, come accennato, mostrano che l'Italia è l'unico tra i Paesi OCSE il cui tasso di crescita, nel 2013, risulterà essere negativo (meno 1,8 Il ritmo della ripresa nelle maggiori economie avanzate è invece aumentato nel secondo trimestre e ci si aspetta che la crescita si manterrà ad un simile ritmo anche nella seconda metà dell'anno. A fronte della nostra situazione specifica, la crescita del secondo trimestre nelle principali economie avanzate nel suo complesso è stata, infatti, più forte del previsto. Gli Stati Uniti hanno continuato a recuperare, nonostante i venti contrari derivanti dal forte consolidamento fiscale. Il PIL dell'area euro, nel secondo trimestre, è cresciuto dopo un periodo di debolezza eccezionale, alla fine del 2012 e al primo trimestre del 2013, mettendo così fine a un periodo di ben sei trimestri di contrazione consecutiva. Nel Regno Unito, la crescita ha ripreso slancio nella prima metà dell'anno. In sintesi, l'Italia rimane l'unica Nazione europea per la quale le buone notizie relative allo stato dell'economia tardano ancora ad arrivare. L'Italia è, quindi, tra le ultime posizioni anche per quanto riguarda la percentuale di crediti bancari inesigibili; solo Irlanda e Grecia si trovano in una situazione peggiore. Anche la *performance* del mercato dell'*export*, tradizionalmente positiva per l'Italia, è risultata in caduta libera negli ultimi anni, soprattutto se confrontata con quella della Germania e dell'Irlanda. Una persistente debolezza degli interventi nelle economie avanzate, successiva alla crisi, ha poi rallentato la crescita del capitale e rischia di frenare la crescita della produttività durante la ripresa. Maggiori progressi verso la rimozione degli ostacoli al commercio e in materia di accordi bilaterali potrebbero contribuire a stimolare la crescita della produttività e dare un nuovo impulso all'aumento del volume degli scambi. Dobbiamo però tutti contribuire affinché ci sia una chiara consapevolezza della situazione che stiamo vivendo. Su questo tema mi limito a rammentare che il 6 agosto scorso, in una intervista rilasciata al termine di un vertice con il *premier* Enrico Letta e i rappresentanti della Banca d'Italia, il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni affermava: «Credo che l'economia entrerà in ripresa, siamo a un punto di svolta del ciclo». Purtroppo le ottimistiche previsioni sono state smentite dagli ultimi dati, che mostrano come l'Italia sia l'unico dei Paesi OCSE il cui tasso di crescita nel 2013 risulterà essere negativo. Peraltro, sono numeri diversi da quelli più positivi a cui si erano riferiti nel mese di luglio sia il Ministro dell'economia sia il Governatore della Banca d'Italia. Infatti, anche la relazione al Parlamento appena presentata dal Governo, ai sensi dell'articolo 10*-bis*, comma 6, della legge di contabilità, attesta questa decrescita, (fino a tutto il secondo trimestre del 2013 indicata come pari a meno 1,7 per cento, ed oggi accertata dall'ISTAT come pari a meno 1,8 cento). Ora, se da un lato è comprensibile che i massimi responsabili della nostra politica economica siano indotti a mandare messaggi di fiducia, dall'altro lato ai messaggi devono seguire i fatti. La diagnosi in proposito è nota: sul piano interno, quello sul quale possiamo provare ad intervenire: si confermano gli antichi e mai risolti problemi della nostra competitività: un eccessivo carico burocratico e fiscale, una bassa efficienza e qualità dei servizi pubblici, tempi della giustizia eccessivamente lunghi. La governabilità faticosamente ottenuta con un accordo di coalizione vasta è un valore da difendere in quanto è la pre-condizione per riavviare la crescita, ma assume un significato concreto solo se saremo in grado di dare soluzioni ai problemi reali del Paese, affrontando e risolvendo le problematiche del mondo del lavoro e delle imprese. Serve un'Italia moderna, più semplice, più leggera; un'Italia dove è facile voler fare impresa e dove la burocrazia non rappresenti mai un ostacolo. Questa è la nostra sfida, e su questa sfida ci misureremo nei prossimi mesi. È iscritta a parlare la senatrice Zanoni. Ne ha facoltà. Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, nel 2012 in Europa gli unici Paesi che hanno presentato un saldo primario positivo sono l'Italia e la Germania. Il *deficit* effettivo o indebitamento netto per l'Italia è stato del 3 per cento, quando invece negli altri Paesi è stato molto più elevato, ad eccezione, naturalmente, della Germania, che presenta un saldo positivo. Nel complesso, tutti i Paesi dell'area hanno migliorato comunque i saldi di bilancio rispetto al 2011, con la Germania in leggero avanzo. Se guardiamo all'indebitamento corrente, cioè alla differenza fra entrate correnti e spesa corrente al netto degli interessi sul debito, l'Italia con il suo avanzo primario rilevante e con un *deficit* di circa il 3 per è quella che ottiene i risultati migliori, dopo, naturalmente, la Germania. Il problema diventa drammatico se guardiamo il rapporto debito-PIL. Il dramma è che chi negli anni passati ha contribuito al disastro finanziario oggi pontifica, vedi la Lega Nord. Nel 2012 abbiamo un aumento di 6 punti percentuali del rapporto debito-PIL e raggiungiamo il 127 per cento rispetto al 120,8 per cento del 2011. Quei sei punti in più valgono, in euro, 80 miliardi. La media dell'area

La pressione tributaria è risultata il 30,1 per cento del PIL e quella fiscale raggiunge il 44 per cento, in aumento rispetto al 2011 dell'1,4 Il rapporto debito-PIL cresce così tanto perché il debito in termini di oneri ci costa molto e, di contro, non abbiamo una crescita del PIL. Esistono anche altri fattori, ma producono effetti minori. Il valore del nostro PIL nel 2012 era pari a circa 1.566 miliardi di euro, con una flessione dello 0,8 per cento rispetto al 2011. Nel 2012 il prodotto interno lordo in Italia ha avuto una variazione negativa del 2,4 per cento, con una previsione di meno 1,3 per cento nel 2013 e un più 0,7 per cento Percentuali che, per quanto riguarda il 2013 e 2014, sono nettamente negative rispetto alle previsioni della media dei Paesi europei e dell'area euro. Con queste previsioni il nostro debito pubblico continuerà naturalmente ad aumentare. La spesa corrente nel 2012 rispetto al PIL aumenta dello 0,7 per cento rispetto al 2011, mentre la spesa nel 2011 era diminuita sensibilmente rispetto al 2010. L'aumento è da imputare alla spesa per le prestazioni sociali e, soprattutto, agli interessi passivi, che nel 2012 sono aumentati di oltre 8 miliardi rispetto al 2011, arrivando alla cifra di oltre 86 miliardi di euro. La previsione nel DEF 2012 per gli interessi era di 2,5 miliardi in meno rispetto al consuntivo. Oggi la spesa corrente si attesta intorno al 48,1 per Credo sia di fondamentale importanza analizzare i dati di previsione con i dati di consuntivo. Gli obiettivi di finanza pubblica che ci eravamo assunti per il 2012 sono stati modificati con numerose manovre finanziarie, quantificabili in circa 60 miliardi di euro. Le manovre correttive sono state necessarie perché le previsioni riguardo il PIL si sono dimostrate ben peggiori di quelle preventivate. a dimostrazione che l'adozione di politiche di bilancio troppo stringenti non favorisce la crescita economica, che è fondamentale per il risanamento delle finanze pubbliche. La politica dell'aumento della pressione fiscale per compensare la caduta del gettito, a seguito della perdita di prodotto interno lordo, non ha portato ai risultati preventivati. Nei fatti, una maggiore imposizione in una fase recessiva porta ad un ulteriore rallentamento dell'economia reale. Le entrate tributarie sono, sì, aumentate, ma sono ben al di sotto degli obiettivi preventivati: 11 miliardi in meno rispetto alla Nota di aggiornamento del DEF di settembre e di quasi 30 miliardi rispetto al DEF 2012. A fronte di un mancato gettito e di una flessione del PIL si è voluto aumentare la pressione fiscale, con conseguenze disastrose rispetto alle previsioni di bilancio. Nel 2012 è stato il mancato conseguimento della previsione delle entrate a far saltare gli obiettivi di saldo. Le manovre di bilancio fra settembre e dicembre 2012, alla luce della flessione nominale del PIL, hanno provocato un forte aumento della pressione fiscale. La Corte dei conti ci dice che, oltre al cedimento delle entrate, sono state prese decisioni che hanno indebolito 1'attività di riscossione, togliendo strumenti operativi a disposizione degli agenti di riscossione e soprattutto ci mette in guardia su «una realtà cui, peraltro, si è andata aggiungendo un'evidenza, non meno preoccupante, che i consuntivi del 2011 non avevano ancora colto pienamente: l'appannamento del ruolo, finora molto rilevante, attribuito dalla politica tributaria all'ampliamento delle basi imponibili e al recupero del gettito sottratto dall'evasione e dall'elusione». Il gettito fiscale è stato inferiore di quasi 90 miliardi rispetto alle stime di inizio legislatura, e questo ha comportato il mancato conseguimento dell'obiettivo di disavanzo. Il consuntivo di legislatura evidenzia, quindi, che la mancata realizzazione del pareggio di bilancio è dovuta alla caduta del gettito fiscale che deriva dalla perdita di prodotto in cui è incorsa l'economia italiana. Nonostante questo, la pressione fiscale è aumentata rispetto alle previsioni di bilancio (43,1 per cento), arrivando alla cifra record del 44 per cento del PIL e la spesa primaria, pur a fronte dei pur a fronte dei forti risparmi conseguiti, è passata dal 43 al 45,6 per cento del PIL. Questo è il dato fondamentale che, a mio avviso, ci viene da questo rendiconto: le previsioni sono state completamente sbagliate e disattese

il dovere di contribuire a rafforzare, a cominciare dalla legge di stabilità che prossimamente il Governo e il Parlamento dovranno esaminare, per dare più forza ed agganciare quella ripresa internazionale che da più parti viene giustamente valorizzata. La seconda osservazione che intendo svolgere riguarda proprio la struttura del rendiconto. Come si è detto già nella relazione, approvare il rendiconto non significa nascondere le criticità che emergono nella sua struttura; piuttosto occorre fare in modo che il rendiconto permetta di evidenziare con più forza il rapporto tra l'allocazione delle risorse e il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione. Questo purtroppo oggi non è facilmente individuabile:

la spesa pubblica ai fini del controllo e di una destinazione più propria e più precisa verso obiettivi di crescita e di sviluppo. Grazie.

del 20 aprile 2012 - che va a farsi benedire e il pareggio di bilancio che si allontana. Crescono le spese, non solo quelle relative al costo del debito pubblico; diminuiscono le entrate: IVA, accise sui carburanti, entrate tributarie. Su una cosa mi è sembrato di capire, ascoltando gli interventi, che siamo tutti d'accordo: bisogna far ripartire l'economia. Questo è l'unico modo per superare questa situazione. Bisogna far crescere il PIL, abbassare il costo del lavoro, creare nuova occupazione, per avere a disposizione nuove risorse libere da destinare ai problemi che sono stati sollevati.

ha toccato alcuni argomenti, ribadendo che vi è una necessità evidente di rendere più intelligibile e trasparente, dal punto di vista della qualità dell'identificazione della spesa, il rendiconto generale dello Stato, trattandosi di un elemento che consente di individuare la responsabilità nella spesa, soprattutto amministrativa. Questo è uno degli elementi strategici di cambio di passo per i prossimi anni i Governi che dovranno impegnarsi su questo versante dovranno comunque portare avanti, in una logica di maggiore efficacia e di continuità. Per quanto concerne l'aspetto relativo all'assestamento, innanzitutto vorrei rappresentare e precisare nuovamente che le variazioni apportate con il provvedimento di assestamento, unitamente alle variazioni di bilancio, riguardano il periodo tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2013; proprio queste determinano il bilancio assestato. A seguito delle suddette variazioni, il saldo netto da finanziare in termini di competenza, approvato con la legge di bilancio 2013, passa da meno 6.185 milioni di euro a meno 31.066 milioni di euro. Larga parte di quel peggioramento del saldo deriva dalle variazioni di bilancio adottate nel periodo gennaio-maggio 2013, con effetti negativi complessivi per 16.586 milioni di euro. Quelle variazioni sono connesse all'attuazione del decreto-legge n. 35, per 10,5 miliardi di euro; all'assegnazione di 2 miliardi di euro in favore del Monte dei Paschi di Siena, ai sensi del decreto-legge all'attribuzione delle risorse finanziarie rivenienti dalla privatizzazione SACE-SIMEST. Si tratta di provvedimenti che autorizzavano spese coperte con emissioni di titoli del debito pubblico, quindi non compensate.

le variazioni di bilancio connesse all'assestamento 2013 riguardano soprattutto puntuali scelte di ordine politico, che hanno che hanno affrontato situazioni di emergenza che si sono riverberate, poi, su questa necessità di intervento di assestamento. Esse non derivano, quindi, semplicemente da un andamento poco attento delle dinamiche connesse al bilancio dello Stato. Per quanto riguarda sempre l'assestamento del 2013, vi è un peggioramento del saldo netto da finanziare in termini di competenza di 9,9 miliardi di euro, euro, dovuto complessivamente ad un'altra serie di motivazioni - che è giusto ribadire - che hanno evidentemente dei contenuti prettamente politici. Per quanto concerne le entrate finali, si è tenuto conto ovviamente del quadro macroeconomico definito nel DEF di aprile 2013, che scontava già la diminuzione delle entrate tributarie,

il gettito dei primi sette mesi del 2013, complessivamente, dimostra un elemento di crescita addirittura dell'1,2 per cento, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: ovvero risulta superiore al tasso di crescita Insomma, l'assestamento di bilancio va letto non solo, ovviamente, nelle parti che devono essere progressivamente migliorate dalle azioni di Governo che dovranno essere adottate nei prossimi mesi, ma anche in una chiave positiva. Non tutti gli elementi in materia di entrata e di gestione delle entrate, infatti, sono stati negativi: abbiamo una serie di dati che ci hanno consentito oggettivamente di restare in piedi. Mi permetto di dire che anche le entrate extratributarie hanno registrato un aumento di 2.088 milioni di euro, dovuti in gran parte alla previsione del riversamento, nell'entrata del bilancio statale, delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali intestate all'Azienda dei monopoli di Stato. Le spese, nel complesso, si riducono di 2 miliardi e mezzo, principalmente per i minori trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di adeguare gli stanziamenti iniziali all'effettivo livello delle entrate tributarie direttamente riscosse. Anche la spesa per interessi registra una diminuzione interessante, che è un elemento che possiamo considerare anche un valore, con buona probabilità, per i prossimi mesi. In ordine alle variazioni positive sulle spese connesse con il funzionamento delle amministrazioni, si devono anche segnalare elementi di efficienza che riguardano

di sostegno ai soggetti deboli, le risorse che vengono trasferite alle Regioni, insomma quella quantità di risorse molto importante, ma difficilmente comprimibile senza intaccare la qualità servizi. Per quanto riguarda le variazioni proposte, è giusto sottolineare che tutti questi interventi non determinano impatti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno statale, quindi complessivamente non vanno a peggiorare ‑ come è stato ricordato da qualcuno ‑ un quadro di finanza pubblica che, altrimenti, sembra in qualche modo fuori controllo. La finanza pubblica non è fuori controllo:

dei debiti della pubblica amministrazione. Più in generale, dobbiamo anche riconoscere che ci sono stati alcuni passaggi che riguardano le integrazioni delle dotazioni di cassa, il rimborso di prestiti relativo in particolar modo

Grazie.

la qualità delle coperture è un elemento fondamentale. Da questo punto di vista credo che la certezza, insieme alla qualità, sia la sfida che attende non solo il Governo, ma anche il Parlamento.

più eque rispetto a quelle tradizionalmente utilizzate, ma che possano anche essere accettate in sede europea, l'altro importante aspetto che molto spesso viene trascurato ma che rappresenta per noi un punto di riferimento che non possiamo evitare

una volta conclusa la votazione degli articoli del rendiconto, si passerà direttamente all'esame degli articoli dell'assestamento. Seguiranno poi le dichiarazioni di voto congiunte e avranno quindi luogo le due votazioni con il sistema elettronico. Procediamo dunque all'esame degli articoli del disegno di legge n. 888.

continuamente dei messaggi. Ritengo che, forse, nel rispetto di quest'Aula e dei senatori che stanno partecipando numerosi a questi lavori, lei debba assumere un atteggiamento sicuramente più rispettoso.

comma 3, della legge di contabilità, con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi della stessa missione di spesa ed esclusivamente per le spese rimodulabili derivanti da fattori legislativi. Pertanto, conformemente a quanto già stabilito nel corso dell'esame in sede referente, la Presidenza dichiara inammissibili gli emendamenti 1.Tab.2.1, 1.Tab.2.2, 1.Tab2.3,

C'è chi giura di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno prescindendo da etnie, religione, nazionalità, condizione sociale ed ideologia politica; di assistere...

ringrazio, signor Presidente. Sono veramente molto frastornato da questo atteggiamento. Inizio da capo, signor Presidente, semplicemente perché non sto parlando di calcio, né di sport, né di qualche altro argomento un po' più frivolo, ma sto parlando di una questione legata ad un dramma, a qualcosa che è stato considerato un orrore. dicevo, signor Presidente, nella vita si giura su molte cose e per tante cose: «Giuro di curare ogni paziente, con eguale scrupolo ed impegno, prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale ed ideologia politica; di prestare assistenza d'urgenza a chi ne ha bisogno». Forte questo giuramento e di questa convinzione, domenica sera nel comune di Chiuduno, in Provincia di Bergamo, Eleonora Cantamessa, uno splendido medico di 44 anni, transitando in auto con un amico si è fermata per prestare aiuto a una persona sconosciuta, a un uomo indiano ferito in una rissa. Un'auto con quattro connazionali del ferito - i suoi aggressori - ha falciato entrambi, probabilmente con lo scopo (su questo sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri) di «finire» definitivamente l'uomo da loro stessi accoltellato. Signor Presidente, un angelo è morto per aver portato fede a quel giuramento: ha perso la vita perché il suo cuore era troppo grande e troppo grande era la sua generosità, e quella generosità non aveva limiti. Era molto brava, semplice, dolce, disponibile e generosa; era fatta così, e non poteva non fermarsi. Non ha mai chiuso la porta in faccia a nessuno. Questi sono tra i commenti che più hanno accompagnato le ultime ore. Chi la conosceva bene ne ha apprezzato la vita in questi 44 anni: una ragazza che aveva dato la sua vita per una professione così importante. Il bilancio di quello che sembra essere a tutti gli effetti un sanguinoso regolamento di conti tra immigrati è di due morti e otto persone ferite. si è sempre molto perplessi quando si parla di questi casi, perché si viene accusati di razzismo e di facile demagogia;

noi come Gruppo abbiamo assolutamente preso in considerazione tutti i lati di questo orrore, di quello che è stato considerato un fatto da *Far West*, perché è stata distrutta una famiglia.

Signor Presidente, mi dispiace dover tornare sull'argomento, ma mi rivolgo ancora cortesemente al Presidente del Senato per ricordare che il Governo italiano ha firmato

perché siamo ancora una Repubblica parlamentare. Il Parlamento è la sede della sovranità popolare ed è inaccettabile che accordi di questa rilevanza non siano conosciuti dai parlamentari, i quali possono darne un giudizio, positivo o negativo che sia. Tuttavia, prima di dare un giudizio, sarà bene conoscere il contenuto dell'accordo, che - ripeto - è già stato firmato dal ministro Delrio e dal presidente Durnwalder, e che è oggetto di polemiche da campagna elettorale.

Signor Presidente, poco fa il collega Consiglio ha fatto riferimento alla dottoressa drammaticamente e tragicamente ammazzata nel

Paola Labriola, una psichiatra brava e amatissima dai suoi pazienti, nell'esercizio della sua attività professionale presso il Centro di igiene mentale del quartiere Libertà a Bari, è stata ammazzata, uccisa da 30 coltellate, inferte che con violenza efferata un assistito nell'addome fino a farla stramazzare a terra senza vita. La città è rimasta attonita. Il Paese si è interrogato su questa striscia di sangue che si allunga inesorabilmente fino a lambire le porte delle istituzioni. Oggi, dobbiamo chiederci nelle sedi competenti, nelle Aule del Parlamento, se è possibile che in un Paese civile si finisca col morire di lavoro. Questa collega, questa dottoressa, infatti, questo medico, è morta ammazzata servendo lo Stato, servendo i suoi pazienti, prestando fede al giuramento di Ippocrate. Signor Presidente, Signor Presidente, affido alle valutazioni di quest'Aula la drammatica circostanza di questo e dell'altro efferato delitto, perché, indubbiamente, va fatta una riflessione seria compulsando adeguatamente il Ministro della salute, ma anche i Ministri dell'interno e del lavoro. Non abbiamo ricette magiche e non consentiremo a nessuno di fare alcun tipo di speculazione su queste morti. Il problema è drammaticamente inquietante, interroga le nostre coscienze. C'è l'evidente necessità di ripensare i sistemi di sicurezza

Probabilmente la questione può essere affrontata con un intervento che, lungi dall'ipotizzare una militarizzazione dei presidi sanitari, porti però ad introdurre sistemi che, anche attraverso l'inserimento nelle strutture pubbliche, possano consentire lo svolgimento regolare dell'attività, garantendo di più e meglio la tutela della vita di chi all'interno di quelle strutture opera e a quelle strutture si rivolge. Questo è il monito che ci viene, perché non saranno sufficienti le giornate di lutto proclamate dai sindaci né saranno sufficienti le migliaia di persone intervenute ai funerali, con parole toccanti dell'arcivescovo, a tacitare le nostre coscienze. Dobbiamo fare in modo che queste tragedie ci spingano in maniera concreta verso una soluzione che sia la più adeguata e la più idonea. Il Paese l'attende, così come